L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

nella seduta antimeridiana sono stati accolti gli ordini del giorno su cui i relatori ed il rappresentante del Governo avevano espresso parere favorevole. Passiamo quindi all'esame degli ordini del giorno, su cui i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

decretata dall'Unione europea, che ha come scopo la protezione delle navi del programma alimentare destinato agli sfollati in Somalia. La Somalia, contrariamente a quanto si possa pensare, non è un territorio interamente iscrivibile tra i cosiddetti Stati falliti: nel Nord del Paese esiste una Regione, che si chiama Somaliland, dove

di uno Stato che non è riconosciuto da nessuno, anche se gode di uno *status* speciale all'interno dell'Unione africana. L'ordine del giorno G200 intendeva porre all'attenzione del Governo di stabilire se non altro un rapporto di collaborazione con il Somaliland, visto e considerato che in passato la Francia ha utilizzato il porto di Berbera, che ne è l'ex capitale, per stazionarvi

al subappalto di determinate funzioni che spesso i Governi si trovano a dover accordare a imprese private per attività di logistica, ma sempre più spesso - ahinoi - anche pienamente militari.

i servizi ricordati (funzioni militari e anche logistiche), sia comunque di impegnarsi a mantenere il massimo rispetto dei principi enunciati dai quattro Paesi nostri partners

Come si può notare dalle tre pagine di "considerando", sono ormai tre anni e mezzo, quasi quattro che la comunità internazionale si interroga sulla possibilità

per fini medici e far diventare l'Afghanistan uno dei quattro o cinque Paesi che forniscono questa materia prima per la produzione di morfina e codeina. Esistono - e lei, signora Presidente, lo sa meglio di altri, visto che che nel settembre 2005 era a capo della missione dell'Unione europea che monitorava le elezioni parlamentari in quel Paese - una serie di delibere formali in tal senso, sia del Parlamento europeo, due volte è tornato sulla questione, sia del Parlamento italiano della scorsa legislatura che alla Camera dei deputati, con un ordine del giorno prima e una mozione poi, ha chiesto all'Italia, di concerto con i partner europei, di prendere in considerazione il lancio di progetti pilota per la produzione di papavero, e non di oppio, per farne analgesici da distribuire poi, attraverso un apposito fondo delle Nazioni Unite, ai Paesi poveri o in via di sviluppo che non hanno accesso minimo a questo tipo di medicine per la cura del dolore. proprio perché non aiuta nascondere la testa sotto la terra tutte le volte che parliamo di Afghanistan e, quindi, far finta che non esista

Nulla osta a che questa riga possa essere soppressa se il Governo dovesse far proprio il parere del relatore e, quindi, accogliere come raccomandazione la

Il Governo è disposto ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G203 limitatamente alla prima parte del dispositivo, cioè sino alle

Si chiede inoltre di ampliare la relazione semestrale che il Ministero deve presentare alle Camere, compresa quella scorsa del 15 novembre che, a nostro parere, risulta troppo generica.

il Governo: a riferire alle Camere, preventivamente alla predisposizione di progetti di cooperazione allo sviluppo che si intendono avviare avvalendosi della collaborazione di personale estraneo alla pubblica amministrazione, circa la natura degli stessi progetti, precisandone le finalità, l'organizzazione, il costo e la durata complessiva, evidenziando altresì le ragioni per le quali non è possibile provvedere alla svolgimento degli stessi con il personale in servizio;

studi e incarichi di consulenza, stabilendo che le stesse non potessero essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2004. Il Ministero, con quel comma 3, può avvalersi di tale deroga per stipulare anche con enti e organizzazioni specializzate contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Quindi, si richiede di illustrare preventivamente la conclusione dei contratti la natura dei progetti di consulenza e di precisarne le finalità, l'organizzazione, il costo e la durata complessiva. Questo per il contenimento dei costi. L'Italia dei Valori ritiene che il comma in questione sia troppo generico nella formulazione e lasci eccessiva discrezionalità finanziaria e di gestione al Ministero. E continuiamo a parlare di costi della politica.

Infatti, derogare alla norma tetto della finanziaria 2006, finalizzata alla razionalizzazione delle risorse nonché alla limitazione degli sprechi che spesso si annidano proprio in consulenze e prestazioni occasionali ben retribuite, significa negare tutta quella ricerca dell'efficienza amministrativa che questo Governo ha tanto pubblicizzato con l'opinione pubblica (dai fannulloni, al rigore in finanziaria),

che verrà presentata al Parlamento a breve, maggiori informazioni concernenti i risultati raggiunti, l'efficacia degli interventi e il completamento degli obiettivi fissati, così come stabilito dall'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231. È la «Relazione sulla partecipazione

tale possibilità. Nel corso della discussione è stata oggetto di emendamenti presentati in Commissione anche la proposta di porre in capo al Governo l'obbligo di presentare un documento consuntivo dello *status quo* delle missioni all'estero 40 giorni prima del finanziamento delle stesse e di utilizzare questo documento come base per proporre linee e principi da seguire nel decreto di rifinanziamento. quindi, sullo spirito della proposta, ritenendo che, ogni qualvolta si discute di missioni nelle quali sono impegnati i nostri militari, sia necessario arrivare a formulare una valutazione politica dell'impegno estero. Credo che un apprezzamento di carattere sostanziale solo economico, come avviene con il decreto di proroga, non sia sufficiente. Ricordo che dalla lettura del documento del Senato recante «Relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso», concernente il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2008, presentato dal ministro Frattini in data 15 novembre 2008, si evince che la previsione contenuta nell'articolo 14 della legge menzionata non è stata trattata con la dovuta attenzione. altre parti della relazione - ripeto, mi riferisco alla relazione firmata dal Governo Berlusconi del 2003 - appaiono sommarie ed incomplete nello spirito generale e si riscontra una mera descrizione una mera descrizione di attività portate avanti dai contingenti, senza nessuna comparazione tra ciò che ci si era riproposti di conseguire con le missioni e ciò che in effetti è stato conseguito. Mi riferisco alla missione a Cipro (anche il collega Perduca questa mattina ne ha fatto

In tal senso, il Gruppo dell'Italia dei Valori chiede di inserire nella Relazione concernente il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e che sarà presentata al Parlamento a breve, maggiori informazioni riguardanti l'effettività dei risultati raggiunti. Nell'ultima relazione sono stati trascurati. ritengo utile utilizzare lo strumento della relazione semestrale, già stabilito nel nostro ordinamento, piuttosto che introdurre un nuovo strumento che è la legge quadro sulle missioni internazionali, la quale presenta tra l'altro un'eccessiva rigidità nella trattazione di una materia che è invece sensibile agli eventi di attualità. Lo strumento della relazione potrebbe magari essere potenziato introducendo una disposizione che vincoli il Governo a seguire nella predisposizione del decreto di rifinanziamento gli orientamenti emersi nella discussione parlamentare sulla relazione. Tale momento di dibattito, se fatto su un testo completo ed esaustivo, come sancisce la legge n. 231, potrebbe rappresentare l'*input* per avviare una discussione sullo stato delle nostre missioni all'estero e sulle ipotesi per una loro ristrutturazione. Quindi, vi chiedo

desidero rispondere. Senatore Pedica, io ho seguito con attenzione i suoi commenti e non le nascondo che su alcune tematiche, dal punto di vista personale, ho memoria di quanto alcuni parlamentari dell'attuale maggioranza hanno detto e fatto nel corso di precedenti legislature.

Come i colleghi sanno perfettamente, esiste una serie di patologie riscontrate tra il personale che rientra dalle missioni all'estero.

nella determinazione degli oneri ordinari.

al Governo libanese gli strumenti che abbiamo impiegato: quindi in parte, lo ripeto, devo considerare queste attività già spesate negli oneri ordinari. relativo all'attività di educazione al rischio mine a favore della popolazione civile - in particolare, e ancora una volta, se parliamo di mine e di *clusters bomb* in relazione al Libano - il Governo fa presente che queste attività potrebbero essere assegnate ai comandanti locali

un'attività molto interessante che vede per la prima volta un'intensa collaborazione tra le ONG e le nostre Forze armate, con un protocollo d'intesa che prevede anche le modalità di suddivisione dei ruoli.

per complessivamente 808.385.522 euro per l'anno 2009 e 250.000 a decorrere dall'anno 2010. Nonostante il summenzionato articolo 7, si riferisca in generale agli oneri per l'anno 2009, il calcolo che li vede quantificati in 808.135.522 attiene quasi totalmente alla proroga delle missioni internazionali limitatamente sino al 30 giugno 2009. Rammento quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007, che autorizza per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 1 miliardo per la partecipazione alle missioni internazionali di pace ed istituisce a tale scopo un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Quindi, al netto dei fondi utilizzati nel presente disegno di legge per il finanziamento delle missioni attinenti al primo semestre 2009, i fondi stanziati dalla legge finanziaria 2007 per coprire gli oneri di spesa che interessano il periodo 30 giugno 2009 - 31 dicembre dicembre 2009 sono quantificati in poco più di 190 milioni di euro. Ritenendo quindi reale il rischio che, per il secondo semestre 2009, non sussistano fondi sufficienti a garantire la proroga delle summenzionate missioni, si vuole impegnare il Governo a valutare il pericolo illustrato e contestualmente ad indicare alle Camere quali fondi alternativi eventualmente pensa di poter utilizzare.

la difesa*. Non posso accogliere questo ordine del giorno per il semplice fatto che non nutro le stesse preoccupazioni del presentatore. Quindi, illustrerò la motivazione per cui non lo accolgo e probabilmente riuscirò anche a togliere alcuni dei dubbi che i presentatori hanno avanzato.

a delle manutenzioni straordinarie in relazione all'impiego dei mezzi in teatro. Questa è la ragione per cui quel fondo, che era stato costruito seguendo un'altra logica, è evidentemente non capiente. capiente. Nell'emanazione di tale decreto, in sede di Consiglio dei ministri (da questo punto di vista il Governo non ha difficoltà a confermarlo), è stata comunque assicurata la copertura degli oneri semestrali, che saranno pari a circa 700 milioni nel secondo semestre, impiegando ovviamente altri fondi presenti in finanziaria, o direttamente o attraverso una nuova alimentazione. La ragione per cui non c'è capienza deriva quindi proprio dalla modifica concettuale delle spese che vengono da questo punto di vista il Governo può serenamente confermare la volontà di mantenere il cosiddetto livello di ambizione in relazione alle nostre missioni all'estero, anche se ciò localmente può comportare delle modifiche, perché il livello di ambizione e di impegno non è ovviamente esclusivamente legato al numero di soldati che partecipano ad una missione o ai soldi che vengono spesi, ma è un concetto più ampio. il Governo si impegna a garantire il finanziamento anche per i restanti sei mesi, anche se è perfettamente a conoscenza del fatto che ciò avverrà attraverso quel fondo che è stato costruito secondo una logica diversa. Quindi, formalmente, come vede, non posso accettare questo ordine del giorno, ma il Governo ha già sostanzialmente provveduto ad evitare che le preoccupazioni da lei espresse si possano concretizzare.

Signora Presidente, colleghi senatori, l'Aula del Senato è chiamata a votare nuovamente, a distanza di poco tempo, la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali. È evidente che non ci sono dubbi sul nostro voto a favore di questo provvedimento, di quello che riteniamo cioè un dovere nei confronti dei nostri soldati, al quale non ci dobbiamo, né ci vogliamo, sottrarre. A loro, ancora una volta, va il nostro profondo senso di rispetto e di riconoscenza, perché con alto senso dello Stato e coraggio portano aiuto alle popolazioni civili, in situazioni spesso di estrema difficoltà e delicatezza, in operazioni di *peace keeping* molto dispendiose sotto il profilo degli uomini, dei mezzi e delle capacità da mettere in campo. Per tali motivi vorremmo che questo non fosse un appuntamento burocratico, cadenzato in pochi mesi, ma che si possa avviare una seria programmazione per dare più certezze ai nostri soldati. In questo senso, non giovano di certo i tagli predisposti ai fondi per la difesa, lontani dallo standard che la NATO ci chiede per rendere affidabile il nostro sistema difensivo. Nel disegno di legge è illustrato, con la necessaria dovizia di particolari, il grande lavoro che i nostri militari stanno svolgendo in ogni parte del mondo e che oggi siamo chiamati a rinnovare: le iniziative di cooperazione in Afghanistan, in Iraq, in Libano, gli interventi per le esigenze di prima necessità delle popolazioni locali di regioni quali i Balcani, il sostegno alla ricostruzione, alla pacificazione, alla stabilizzazione politica di aree in bilico tante parti del mondo. L'Afghanistan appare certamente lo scenario più ricco di avversità. Per stessa recente ammissione del ministro La Russa, siamo di fronte ad una missione pericolosissima, in un clima che, se anche recentemente non sta interessando le cronache dei giornali, si sta facendo di giorno in giorno più pesante. A fronte di un impegno delle truppe italiane a contatto con la popolazione civile, sempre teso alla ricostruzione, i talebani stanno rispondendo con attentati, ordigni esplosivi per le strade, lanci di razzi. Negli ultimi due mesi si sono verificati ben trenta tentativi di attacco nei confronti dei soldati italiani. Il nostro contingente - ci fa sapere lo stesso Ministro - non aumenterà oltre i 2.800 soldati, anche se, qualche ora fa, il Ministro degli esteri ha ventilato la possibilità di un contingente aggiuntivo di circa 200-250 uomini per il periodo di svolgimento delle elezioni presidenziali. Soldati ai quali, in ogni caso, spetterà l'arduo compito di limitare gli atti di terrorismo, di garantire libere elezioni, ma anche di bloccare le attività illegali che arricchiscono i talebani; esempio, al commercio di oppio, di cui l'Afghanistan resta, nonostante gli sforzi internazionali, il maggior produttore mondiale. In Libano la situazione appare molto più complessa sotto il profilo politico. Esiste una forza di interposizione UNIFIL, che nacque - lo ricordiamo - anche grazie a un forte impegno congiunto di maggioranza e opposizione nell'agosto 2006, per arginare la guerra tra Israele e i miliziani di Hezbollah. Oggi il Partito di Dio è ancora forte, minaccia con i suoi razzi il confine con Israele e ha insanguinato il Paese con una lunga catena di attentati. Le prossime elezioni di giugno saranno decisive per capire a chi i libanesi daranno fiducia, le conseguenti alleanze del Paese e i rapporti con le vicine Iran e Siria. Restano i rischi per una missione di interposizione che si pone di fatto come cuscinetto di divisione e che quindi riveste grande importanza per la stabilizzazione di tutto lo scacchiere mediorientale, anche se sono evidenti i limiti della nostra interposizione. Nei Balcani, altro punto nodale, la situazione appare congelata, ma in realtà è in grande fermento. C'è da registrare la forte instabilità della Bosnia, ma soprattutto l'indipendenza del Kosovo, che resta un capitolo ancora non chiuso e che rischia di trascendere in scontri di stampo ultranazionalistico, etnico e religioso. La stabilità dei Balcani, vista la sua posizione geografica, deve essere il prima possibile un punto fermo per il nostro Paese e per tutta l'Europa, specie per il rischio che una nuova ondata di profughi da quelle zone possa interessare proprio l'Italia. Tra le altre operazioni che oggi rifinanziamo certamente citiamo quelle per la ricostruzione dell'Iraq, Paese nel quale resta comunque di altissimo profilo il nostro impegno; e poi un impegno che va dalla Georgia, all'Albania, dal Congo a Hebron e Rafah, contro il fenomeno della pirateria sulle coste della Somalia, per la cooperazione contro l'immigrazione clandestina in Libia, di cui molto si è parlato in quest'Aula nei giorni scorsi, grazie all'aiuto della Guardia di finanza e senza dimenticare il contributo di Polizia e Carabinieri per addestrare la polizia locale e renderla quindi pienamente autonoma. Particolarmente significativo, poi, sotto il profilo umanitario, ci pare il nostro prossimo impegno in Darfur, dove da anni viene perpetrato un genocidio dimenticato quasi del tutto dai mezzi di informazione, un nuovo Olocausto di fronte al quale si vorrebbe chiudere gli occhi. L'Italia sarà presente, seppur limitatamente alle sue potenzialità, con personale militare alla missione UNAMID, che raggruppa forze delle Nazioni Unite e dell'Unione africana. Ci interroghiamo semmai su una possibile razionalizzazione delle risorse e degli uomini, per esempio in scenari come quello albanese, dove da molti anni la situazione dell'immigrazione clandestina appare normalizzata e dove quindi il nostro impegno può essere, crediamo, limitato e le forze dislocate in altri luoghi più a rischio. Signora Presidente, colleghi senatori, i nostri soldati impegnati in ogni parte del mondo oggi ci chiedono di metterli in condizione di fare il proprio dovere: portare la pace, aiutare le popolazioni in difficoltà, ricostruire laddove una guerra ha distrutto, garantire lo svolgimento di una vita democratica. Lo faremo, convinti della necessità che le nostre Forze armate abbiano il riconoscimento e il sostegno che meritano, ben maggiore di quello che hanno oggi, perché venga valorizzata sempre più la funzione fondamentale che svolgono: portare il Tricolore nelle parti più difficili del mondo, rappresentando con coraggio e abnegazione l'Italia e i suoi migliori valori.

l'Italia dei Valori ha preso posizioni caratterizzate da senso di responsabilità istituzionale, da attenzione alle esigenze dei militari impegnati all'estero, anche da diversi anni, nonché da un approccio dialogante e aperto con la maggioranza di Governo. Delle missioni all'estero il tratto che osserviamo con più favore come Italia dei Valori è quello del multilateralismo. In un contesto internazionale complesso, in cui la singola forza di ogni Stato nazionale impallidisce rispetto alle organizzazioni criminali sopranazionali ed in cui ogni aspetto della vita pubblica, da quello economico a quello politico, è intimamente legato alle vicende estere, confermare un impegno multilaterale è l'unica via per poter esercitare un ruolo di primo piano. Si invita, quindi, il Governo a continuare sulla linea che caratterizza la nostra politica estera, ribadendo, con mezzi e finanze, la partecipazione italiana a missioni ONU, a operazioni NATO, agli impegni dell'Unione europea e alle attività OSCE. È di poche ore fa la notizia che la Repubblica Ceca ha ratificato, dopo molti rinvii, il Trattato di Lisbona, che, come ricorderete, prevede un rafforzamento della politica estera comunitaria, dà uno *status* giuridico autonomo all'Unione europea nelle relazioni internazionali e rivaluta la figura dell'Alto rappresentante per la PESD. Dunque, anche con tale piccolo passo ulteriore, ci si avvia verso un'epoca in cui o si è multilaterali ed europei o non lo si è. Per tali motivi, come ho rilevato in discussione generale, quando l'Italia conclude, come ha fatto con la Libia, trattati bilaterali (anzi unilaterali se si considera quanto il nostro Paese dà e quanto riceve dalla Libia) l'Italia dei Valori è e sarà fortemente critica ed esprimerà i suoi dubbi sull'utilizzo di risorse per sancire tale antidemocratica alleanza, come si è fatto al comma 25 dell'articolo 3 dell'Atto Senato n. 1334 oggi in esame. E critica sarà di nuovo, lo anticipo colleghi, la nostra posizione in ordine alla discussione in Aula, domani mattina, relativamente all'ultimo accordo frutto di una volontà personalistica del *Premier*, ossia quello di una cooperazione in materia giudiziaria e di polizia concluso con la Russia. Tuttavia, quando si tratta di approvare provvedimenti come quello di oggi, in cui lo spirito generale va nel senso di una *partnership* europea e di una condivisione di oneri ed onori con gli altri Paesi, non possiamo che essere d'accordo. Rimangono però alcune ombre sul provvedimento, che riguardano principalmente la mancanza da parte del Governo di un'analisi globale della nostra linea di politica estera. Penso, ad esempio, alla situazione afgana. Sempre dalle agenzie di questa mattina, si apprende che l'Italia sta valutando l'invio di rinforzi, per qualche centinaio di uomini, con l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle elezioni presidenziali afgane del prossimo 20 agosto. Lo ha annunciato il ministro Frattini, che si trova alla base dei militari italiani ad Herat, nell'Ovest dell'Afghanistan. Tale annuncio porta chiaramente con sé un messaggio circa l'estrema fluidità delle condizioni e l'instabilità della regione. Pertanto, oltre che confermare il nostro impegno nell'area, come si fa con il decreto-legge di proroga delle missioni, ed annunciare un aumento delle forze per le elezioni ad Herat, sarebbe utile che il Ministro venisse in Aula e prevedesse un momento di confronto più generale sullo stato del Paese afgano, sui risultati conseguiti dai nostri soldati, sulla necessità di riformulare la missione, magari concentrandola di più su iniziative economiche che contrastino l'economia illegale degli oppiacei, base di finanziamento dei terroristi. La necessità di condurre un confronto di ampio respiro fra Governo, Ministero degli esteri e della difesa e Parlamento, si evidenzia anche su altri punti deboli del disegno di legge, quelli in cui si rifinanziano missioni composte da pochissimi uomini, come a Haiti, Cipro o Malta, sulla cui reale effettività è lecito nutrire dei dubbi. Anche sulla crisi nella Striscia di Gaza, in cui i rifugiati e la popolazione civile versano in condizioni drammatiche, sarebbe importante - ed è già stato più volte richiesto - un confronto volto a definire possibili iniziative future, che risultano sempre più utili ora che anche il Governo israeliano si caratterizza per un'estrema debolezza. Solo oggi il presidente israeliano Shimon Peres inizierà le consultazioni per decidere a chi assegnare l'incarico di formare il nuovo Governo dopo le elezioni del 10 febbraio. Da quanto detto fino ad ora, si desume chiaramente che lo strumento della decretazione d'urgenza sulla proroga delle missioni internazionali e sul loro rifinanziamento non è sufficiente per esaurire l'impegno di tutti sulla politica internazionale. Si adoperino, dunque, gli strumenti che l'ordinamento prevede. Tra di essi è importante citare la relazione che è stata oggetto dell'ordine del giorno dell'Italia dei Valori, purtroppo non letta e non compresa dal Governo, come avrò tra breve. Oppure se ne inventino di nuovi, basta che si arrivi ad una consultazione complessiva su ciò che l'Italia fa al di fuori dei suoi confini e su come lo fa. Ai rilievi mossi sinora si associano, poi, quelli di carattere economico circa la copertura finanziaria del provvedimento, che impiega praticamente tutte le risorse del 2009 per coprire solo - lo sottolineo - i primi sei mesi dell'anno. Spero che, anche stimolati dalle nostre riflessioni, si possa fare chiarezza sul punto. Mi è dispiaciuto che il Governo

Anche il Partito Democratico in questo momento non ha letto questo impegno e credo non abbia letto quello che nel 2003 è stato votato dal centrodestra. Questo è un atto di irresponsabilità da parte di un Governo che fa le leggi

di ferma lotta quando si propongono decreti e linee politiche incostituzionali o irragionevoli. Di cooperazione, di proposta costruttiva, però, di dialogo aperto, quando si trattano provvedimenti che mirano a mantenere l'Italia un Paese influente e capace di fare la differenza per tanti popoli, per tante sofferenze, per tanti conflitti. Oggi, colleghi,

ruolo di cooperazione. L'Italia dei Valori, nonostante i rilievi mossi, voterà positivamente alla conversione del decreto-legge. L'Italia dei Valori ritiene infatti che la pace e gli sforzi per il raggiungimento di questa, non abbiano colore politico, ma solo il bianco rosso e verde di una Italia bella, che si impegna per garantire condizioni democratiche e pacifiche in tanti Paesi, in tante realtà.

il decreto-legge di proroga delle missioni militari internazionali delle nostre Forze armate è stato varato dal Consiglio dei ministri il 18 dicembre; è stato quindi varato in anticipo rispetto a quanto avveniva negli scorsi anni, quando occorreva spesso attendere la metà o la fine di gennaio, e questo per noi è un valore aggiunto e sicuramente fa onore al Ministro e al Governo tutto. Questo è uno dei segnali che, secondo noi, il comparto della Difesa si aspettava e che è stato dato: un netto cambio di marcia, un approccio nuovo ed un rinnovato dinamismo del Governo rispetto alle missioni internazionali gioveranno sicuramente alle nostre Forze armate e a tutti i militari che vi sono impiegati. Tuttavia, questo non è il solo elemento sostanziale di novità che merita di essere esaminato,

dell'entità delle risorse allocate agli interventi, per consentire la prosecuzione di quelli all'estero fino al 30 giugno.

e di altri 32 milioni per la realizzazione delle infrastrutture d'interesse dei militari italiani nuovamente schierati all'estero. L'incremento che si va a delineare è tanto più significativo se si tiene conto del fatto che a luglio sarà difficile realizzare risparmi sulle missioni che risultano ancora in corso, seppure si pensi già agli eventuali tagli che si potrebbero effettuare sul Libano, sulla Bosnia Erzegovina e sul Ciad. In seguito al varo di questo provvedimento oggi all'esame dell'Aula del Senato, crescerà senza dubbio la presenza in Afghanistan: riteniamo che sarà così e - come si era già intuito all'indomani della conclusione della visita a Roma del generale

di partecipare agli sforzi delle Nazioni Unite e dell'Unione africana in Darfur, stanziando 5,5 milioni di euro per permettere a 100 uomini e a due elicotteri la partecipazione

Alla Camera dobbiamo tener presente anche che con opportuni emendamenti si ha avuto cura di inserire disposizioni che permettano ai nostri militari imbarcati di catturare e perseguire adeguatamente coloro che si sono macchiati di questo crimine di pirateria. Colleghi, abbiamo davanti ai nostri occhi forse il provvedimento più importante di politica estera e di sicurezza nazionale di questo semestre del 2009. un disegno di legge in cui si esprime la volontà del nostro Paese di fare la sua parte nella lotta al terrorismo internazionale e al fanatismo religioso, per la creazione di un mondo più stabile e, soprattutto, prevedibile. In conclusione, vorrei inoltre muovere alcune considerazioni e dare un suggerimento al Ministro: come ha già ribadito il mio collega di Gruppo, missione dopo missione, il nostro Paese sta dimostrando con i fatti di essere presente ovunque e di contribuire con grande generosità agli impegni internazionali assunti. Inoltre, le nostre Forze armate, con i loro uomini, non hanno mai occupato nulla nel mondo; anzi, hanno dato tanto, e le affermazioni e le affermazioni che faccio sono supportate da alcuni fatti. L'esempio più lampante è costituito

Dobbiamo prendere atto che tutte le forze politiche hanno cercato, chi in un modo chi in un altro, con alcune diversità, di appoggiare *in toto* le missioni

Grazie, vorrei iniziare a svolgere qualche riflessione muovendo da un'affermazione appena pronunciata dal collega Torri, il quale, ritengo con molto acume politico, ha considerato che quello in discussione questa sera è l'atto più importante di politica estera che un Governo compia nel corso di un anno solare. Ciò che purtroppo contrasta e stride rispetto a questa affermazione così impegnativa è è il risultato del contesto in cui questa discussione, signora Presidente, si sviluppa, una caratterizzazione per niente politica. Il provvedimento che stiamo discutendo sembra essere piuttosto un rendiconto di tipo ragionieristico, anziché una serie di valutazioni di carattere politico. Stiamo parlando di 8.500 uomini per turno (potremmo dire che in tutto sono 40.000) ai quali puntualmente, come rispondendo ad un *refrain* ancestrale, inviamo saluti e baci senza che però a questo tipo di riconoscimento, che può sembrare soltanto di maniera, corrispondano poi i fatti, corrisponda l'impegno. È troppo chiedere al Governo di predisporre un veicolo legislativo che consenta al Parlamento di ragionare di politica relativamente a questi aspetti così importanti? È troppo chiedere che del destino di 40.000 persone si possa parlare con un maggiore senso di responsabilità, senza che questo avvenga in un contesto ripetitivo, scontato, come se piuttosto che parlare di politica parlassimo soltanto di numeri? Eppure i problemi non mancano. Colleghi, per cortesia. per il tramite del suo Vice presidente, nella recente conferenza di Monaco, ha ammesso sostanzialmente il fallimento della politica della della NATO in terra di Afghanistan; ha ammesso che ci vuole più politica, che ci vuole una ricerca maggiore di consenso; ha ammesso che un'intensificazione dell'azione bellica non è ciò di cui c'è bisogno, perché semmai c'è bisogno di interloquire di più e meglio, di aprire fronti di dialogo e di stendere ponti di discussione. Eppure di questo qui oggi non si è parlato. che nel 2008, a causa dei cosiddetti danni collaterali (non poteva essere coniato un più cinico eufemismo),

Non abbiamo sentito parlare, signora Presidente e signori del Governo, neppure della necessità di sollecitare un rapporto nuovo e diverso col Pakistan, con l'Iran, con la Russia, Regioni, Stati, Nazioni dai quali non si può prescindere se si vuole cercare di dare una risposta seria in quella regione così disastrata. Non si è parlato, e ritengo che questo sia l'aspetto politicamente più grave, della schizofrenia di questo Governo, un Governo che predica la sicurezza, che si manifesta e si esprime anche con atteggiamenti marziali accanto ai soldati, che cerca di accreditare l'idea l'idea che sente i problemi di quella categoria, ma che in realtà trascura vergognosamente il comparto della difesa e della sicurezza, ignora i bisogni di quei lavoratori *(Applausi dal *PD)* e cerca di gabbare il popolo italiano con indicazioni di particolare fumosità gabellando per scelte politiche *spot* elettorali, questioni che non hanno niente a che vedere con la soluzione effettiva

ha formalmente manifestato tutta la propria preoccupazione relativamente al fatto che la carenza di fondi e i tagli che sono stati inferti a questo comparto... Forse bisogna raccontare barzellette per essere ascoltati in questo Paese. il generale Camporini, capo di Stato maggiore della Difesa, ha formalmente riconosciuto e dichiarato la mancanza di risorse finanziarie per garantire l'addestramento di queste persone; ha formalmente invitato a stare attenti, perché con questi fondi, con queste disponibilità finanziarie non esistono oggettivamente le condizioni per preparare queste persone alle missioni internazionali. Di questo non si è parlato. Oggi non si è parlato di questo. Si è parlato di altre cose. Si è parlato di tutt'altro, tranne che delle missioni internazionali. Non si è parlato di Gaza. Io trovo sconvolgente Io trovo sconvolgente che con una battuta e, prima ancora, con una dichiarazione del tipo "vorrei ma non posso", sia stato liquidato l'emendamento del Partito Democratico con il quale veniva chiesto a questo Governo di prevedere - e i tempi ci sono, perché il decreto scade il 2 marzo - uno stanziamento - uno stanziamento di 12 milioni di euro per dare una risposta concreta, e non con i lacrimoni, ad un popolo che sta soffrendo. Serra)*. La missione di Gaza, infatti, non è un'invenzione del Partito Democratico, come ritengo non sia stata un'invenzione del ministro Frattini quando un mese fa ne ha riconosciuto l'utilità. E allora perché non accettare questo emendamento? Perché abbarbicarsi all'inviolabilità dei decreti? Di inviolabilità, infatti, si tratta perché, benché esista il tempo per modificarlo

vorremmo sapere per quale ragione non è stato accettato neppure uno dei nostri emendamenti: quello con cui si vorrebbe ridurre la mortalità da parto in Afghanistan; quello con cui si vorrebbero intensificare le vaccinazioni dei bambini che muoiono a grappoli, colpiti dalle malattie endemiche; quelli per il rifinanziamento delle attività di bonifica dalle *clusters bomb*. Qualche mese fa, questa stessa Aula ha solennemente e pomposamente votato una mozione e oggi non si trovano il tempo e la disponibilità di andare oltre un usurato ordine del giorno.

Noi non diremo che questa è una cultura della morte, ma da questo episodio e da queste circostanze così gravi può certamente derivare un invito ad essere più prudenti quando formulate certe considerazioni nei confronti di questa parte politica. Noi voteremo a favore di questo provvedimento perché ci rendiamo conto che esso è necessitato dalle circostanze, ma votiamo contro la politica che il Governo ha attuato ha attuato e ha manifestato in questo preciso contesto. Votiamo contro l'azione del Governo per la sua indisponibilità ad accogliere anche le seppur minime indicazioni

Caro senatore Pedica, se lei intende maramaldeggiare, ritenendo che qui ci sia qualche uomo quasi morto da sfinire, se lei ritiene che il nostro sia un partito in agonia del quale cercare di fare strame con certe lezioni che volentieri rimandiamo al mittente, si sbaglia: il nostro è un partito in piedi. *(Applausi dal Gruppo Signora Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghi senatori,

che pure è emerso da questo dibattito e dal dibattito nelle Commissioni riunite affari esteri e difesa, e che ha visto il Governo sensibile proprio ad un'iniziativa di carattere parlamentare; iniziativa di carattere parlamentare che credo possa essere inquadrata e sostenuta proprio dall'emendamento e dal successivo ordine del giorno che il relatore, senatore Ramponi, ha di questo dibattito è emersa la disponibilità del Governo a fare in modo che nelle prossime circostanze sia meno rituale questo passaggio alle Camere in riferimento a questo specifico tema e sia invece pronto e disponibile il Governo a coinvolgere i due rami del Parlamento su un'importante, fondamentale attività della politica internazionale dell'Italia e della politica della difesa italiana. Io credo che questo aspetto vada sottolineato, avendo presente un fatto importante: le operazioni militari sono uno strumento di progetto politico e quindi bisogna abituarci a discutere sugli obiettivi politici della missione. È necessario parlarne prima, discuterne, capire, conoscere, avere contezza di tutti quegli argomenti che sono stati accolti dal Governo recependo appunto, come dicevo prima, l'ordine del giorno presentato dal senatore Ramponi. Ramponi. È giusto che non si parli di questo tema solamente nel momento in cui il Parlamento viene chiamato alla conversione del decreto. Del resto, lo stesso decreto, nell'articolo di copertura, mostra la portata e l'importanza dell'argomento e di quanto sia giusto e corretto che vi sia un approfondimento. Avere impegnato oltre 800 milioni di euro per sei mesi dà proprio l'immagine chiara di quanto l'Italia voglia essere protagonista, così come lo è, in riferimento alle missioni militari di pace per la crescita e l'organizzazione di quei popoli che hanno bisogno di sostegno ma anche, nello stesso tempo, di quanto l'Italia sia in prima linea a combattere ogni forma di terrorismo,

Grazie, signora Presidente. non hanno potuto che prendere atto della necessità e dell'opportunità di continuare su questa politica internazionale dell'Italia, su questa politica della difesa dell'Italia. dell'Italia. Colleghi senatori, se dovessimo volgere per un attimo uno sguardo all'indietro ci renderemmo conto di come le politiche in tal senso siano cambiate e migliorate.

propenso a far comprendere l'effettivo ruolo che vuole aver l'Italia. Nel momento in cui si parla di affidabilità della nostra Nazione noi siamo felici nel momento in cui si sottolinea il successo per l'ottimo lavoro svolto dai nostri soldati siamo altrettanto felici,

agli impegni previsti in modo specifico da questo decreto che stiamo convertendo. Questa riflessione riguarda il nuovo assetto geopolitico. Siamo di fronte ad un quadro che in questi ultimi anni si è differenziato e dà la possibilità e l'opportunità all'Europa, e all'Italia in modo particolare, di riaffermare con determinazione questa volontà di solidarietà e di presenza nei confronti degli altri popoli.

Grazie,

nostra politica e ad esplicitare questi arricchimenti, che sono impliciti, sono convinto che daremo anche un attestato di maggiore onore agli uomini e alle donne che vestono la divisa fuori dai confini nazionali e a tutti quegli operatori civili che lavorano per la crescita di quei territori. In estrema sintesi, signor

ed esaltare gli intendimenti veri dell'Italia, nei confronti degli altri Paesi, in termini di amicizia e di solidarietà, ma altresì possa reclamare un ruolo più specifico dell'Italia,

a evitare questo brusìo. Chi non è interessato ai lavori può continuare la conversazione fuori dall'Aula. **Discussione

Signora Presidente, già nel 2004 si era ritenuto opportuno accorpare le elezioni amministrative a quelle per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

che per una migliore organizzazione dell'andamento delle lezioni scolastiche, poiché, com'è noto, la maggior parte dei seggi si trova appunto in istituti scolastici. L'ostacolo risiede nel fatto che, mentre la normativa europea prevede che le elezioni si tengano fra il giovedì e la domenica,

in genere si tengono di domenica e nella prima parte della giornata di lunedì. Nel 2002 fu approvata una legge che reintroduceva anche la giornata di lunedì Grazie,

soltanto all'anno 2009. L'articolo 1 si apre infatti con le parole: «Limitatamente all'anno 2009»; questo anche per evitare che con un decreto-legge si vadano a

la principale, ne sono state aggiunte altre, credo altrettanto condivise. All'articolo 2, innanzitutto, ci si occupa del «voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali

inserirla definitivamente nel nostro ordinamento, in modo da evitare nuovi provvedimenti che debbano interessare soltanto una scadenza elettorale. In questo articolo ci si occupa, come ho detto, di coloro che temporaneamente risiedono all'estero per motivi di servizio. Sappiamo bene che, con la cosiddetta legge Tremaglia, approvata a seguito di una riforma della Costituzione, e poi con la legge applicativa approvata alla fine del 2001, si è regolata in modo molto ampliativo la possibilità per i nostri connazionali che risiedono permanentemente all'estero di votare per le elezioni politiche. Andava risolto il problema per i nostri connazionali che temporaneamente risiedono all'estero. Questo si riferisce, soprattutto, alle categorie più numerose che si trovano all'estero per servizio (necessariamente ci si limita a questo tipo di motivazione per la residenza temporanea all'estero).

che si trovano per motivi di servizio all'estero. L'articolo 2 fa in modo che queste categorie di cittadini possano esprimere il loro voto in modo analogo a quanto possono fare i nostri connazionali che risiedono all'estero in via

ma facendoli votare nell'ambito della circoscrizione Estero, affiancandosi pertanto in modo sostanzialmente improprio a coloro che risiedono permanentemente all'estero. Nel 2008 si fece un passo in più, facendo in modo che potessero votare potessero votare all'estero ma come appartenenti ad una delle circoscrizioni italiane: per semplicità, la circoscrizione alla quale appartiene la capitale. In questo provvedimento, tendenzialmente, coloro che voteranno all'estero come italiani temporaneamente ivi residenti voteranno ancora per la circoscrizione di cui fa parte la capitale ma, ove dipendano da da unità militari che hanno sede in altre circoscrizioni, voteranno come se risiedessero o in quanto risiedono - perché spesso è così nella sede del reparto dal quale dipendono, nella maggior parte dei quali casi per l'appunto non è Roma. Vi è quindi un rafforzamento della possibilità di votare per i nostri connazionali all'estero. L'articolo 3 si occupa di un'altra necessità che si prospetta imminente, cioè delle modalità di espressione del voto all'estero per quanto riguarda i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione. È previsto per la prossima primavera il voto su un *referendum* che fu rinviato l'anno scorso

il voto all'estero per gli italiani che vi risiedono temporaneamente, con modalità analoghe a quella prevista dall'articolo 2 per quanto riguarda, invece, il voto per l'elezione dei rappresentanti italiani

negli ultimi anni delle difficoltà di funzionamento. L'articolo 5 riporta una copertura finanziaria che potrebbe a prima vista contrastare con l'intendimento,

la legge non può imporre al Governo di indire le elezioni amministrative insieme a quelle dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, ma solo offrirne la possibilità. Pertanto, non può la Relazione tecnica tener conto di un fatto che è soltanto eventuale. Di conseguenza, qui c'è solo la parte relativa alla maggiore spesa, che peraltro è molto limitata e si riferisce ad

condivisibile e non già di una parte politica o di un'altra, quella di migliorare la possibilità per tutti i nostri cittadini di esprimere il loro voto, sia che si trovino in Italia che all'estero.

Signor Presidente, stiamo dibattendo di un provvedimento di un certo rilievo, sarebbe quindi importante che ci si dedicasse con cura, perché quella elettorale è una materia di assoluta delicatezza sotto il profilo delle libertà, dei diritti di cittadinanza e, in generale, dei grandi temi dello Stato moderno. Permettere a tutti i cittadini di partecipare adeguatamente alla competizione elettorale è un dovere, in una stagione in cui la partecipazione rischia di scemare con una crescente forma di astensionismo. Ecco perché parlare di questo testo ha un peso non rituale. È utile, e certamente di rilievo sotto il profilo, non solo del risparmio (lo ha detto bene il relatore Malan), ma

la necessità di pubblicizzare la scadenza dell'8-9 marzo, vale a dire il termine entro il quale i cittadini comunitari devono chiarire esercitare il proprio voto. Poiché siamo vicini a questa data, sarebbe opportuno che la massima pubblicità venisse garantita ad una scadenza di questa natura. L'altra considerazione che mi pare importante svolgere, rivolgendomi sempre al Governo e al relatore, è relativa ad una maggiore precisione sulla garanzia per i cittadini malati, donne e uomini di diversa età, naturalmente con diritto di voto, di poter gratuitamente usufruire del proprio diritto all'elettorato

la scadenza dell'8 e del 9 marzo da pubblicizzare per i cittadini comunitari e il tema dei cittadini malati. Vorrei aggiungere ancora che, data la natura complessa del provvedimento, si è pensato da parte di diversi

Un primo emendamento - mi riferisco a un dibattito che è già avvenuto in quest'Aula sull'altro provvedimento, in qualche modo omologo e contiguo, sulla soglia elettorale per il Parlamento europeo - attiene al numero di firme necessarie per presentarsi alla scadenza elettorale europea.

per una scadenza così vicina, chi avesse inteso o intendesse presentarsi debba avere per lo meno il vantaggio di dover raccogliere un minor numero di firme. Accanto a questo e in un certo senso della stessa famiglia è l'emendamento sulla possibilità di ottenere un finanziamento laddove si raggiunga la soglia del 2 per cento. Si potrebbe obiettare che vi è un'altra soglia, ormai decisa,

la nostra Aula non dibatta, mi si permetta, signor Presidente, colleghe e colleghi, come se fosse una sorta di pratica da evadere il più presto possibile. È un tema molto importante e tra l'altro è un testo pieno di questioni rilevanti che

emendative, che sono proposte di miglioramento; far sì, insomma, che, anche attraverso la conversione di un decreto-legge apparentemente finalizzato solo all'*election day*, si possa migliorare l'insieme della nostra legislazione.

favore a un provvedimento che stabilisce lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative ed europee. Quindi, il punto di vista del Gruppo sul provvedimento è in sostanza favorevole, soprattutto a causa della motivazione di alleggerimento economico

motivo presentiamo un semplice emendamento, il 4.0.100, che cerca di migliorare la situazione proprio dal punto di vista della dispendiosità. Non è un mistero che, con una modifica legislativa apportata nel 2006 (si tratta del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006), si è stabilito si è stabilito che in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i rimborsi previsti per le elezioni non si sarebbero interrotti con la legislatura in corso, ma sarebbero proseguiti fino alla data di scadenza naturale di questa.

importante perché stabilisce che in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica il versamento delle quote annuali e dei relativi rimborsi è interrotto.

che politico, come nel caso dell'Assemblea regionale, tanto che per potere arrivare all'unificazione del momento elettorale c'era bisogno di una legiferazione in materia e quindi di potersi reimpossessare delle prerogative da parte del Consiglio regionale. Nel prosieguo, la produzione legislativa e anche il modo di prodursi nell'esternazione della decisione rispetto alla scelta dei propri rappresentanti, ha

una maggiore qualità di decisioni e quindi una migliore produzione rispetto agli atti amministrativi propri e non rispetto a quelli prettamente politici che rientrano nella scelta e dunque nel rapporto tra eletto ed elettore. La decisione non è stata scevra da consensi diversi e da altalenanti scelte in proposito: si cominciò già nel 1996, dopo l'innovazione politica dettata dalla scelta del voto e quindi della scelta dei parlamentari attraverso il collegio uninominale e successivamente, quando l'evoluzione l'evoluzione politica aveva determinato questa necessità di risparmio non soltanto economico, alcune Regioni si uniformarono. Il punto di discrimine rispetto al dibattito è stato ritrovato poi nel 2006, di togliere il livello politico della scelta della rappresentanza politico-amministrativa degli enti locali ha trovato il giusto e totale consenso.

si spera che il dibattito consenta una uniformizzazione più elevata, dato che portando il momento elettorale sia al sabato, sia alla domenica avremo una europeizzazione del sistema elettorale. Si viene così, però, a restringere il periodo di meditazione, quello che, come ricordiamo, era stato introdotto dalla legge elettorale del 1948 e che consentiva, attraverso la sospensione dei comizi e della propaganda elettorale tra il venerdì e la domenica, quella meditazione che avrebbe portato, in assenza di ogni pressione, ad una più veritiera, più rispondente, più trasparente, più intimistica espressione della preferenza; si tratta di un tempo bastevole a quello che in quel momento si valutò necessario.

Siamo dell'idea che ormai la velocità della comunicazione, la maturità dell'elettorato, la possibilità che la ricerca del voto possa essere concentrata e ancor più

l'espressione del voto si determina anche, come era previsto nelle precedenti tornate elettorali, di lunedì, in quella giornata si registra una dispersione della capacità di della capacità di lavoro e quindi una disarmonia non soltanto amministrativa per quanto attiene agli enti locali deputati alla raccolta del consenso, alla sua trasmissione ed elaborazione, ma anche una distonia con le esigenze del mondo del lavoro, che il lunedì si produce in attività del tutto diversa che non in quella importantissima dell'espressione del voto e quindi della garanzia di una democrazia. che il Governo e il relatore abbiano evidenziato che la disposizione non consente un ricevimento nel nostro ordinamento futuribile,

che la modifica venga ad essere perimetrata temporalmente soltanto a questa tornata elettorale: quando si dice, infatti, per il 2009, si intende soltanto per quella tornata elettorale. Un'altra osservazione è data da fare:

uno dei motivi per cui ci troviamo assolutamente d'accordo con il provvedimento.

riguardanti il rinnovo degli organismi delle autonomie locali abbia anche una specifica rilevanza politica e civile. Se dovessimo ricominciare la storia delle elezioni nel nostro Paese e, in particolare, dell'espressione del diritto di voto, che è strettamente connesso con i diritti di di cittadinanza, sin dallo Statuto del 1848, potremmo rilevare che queste consultazioni introducono il cittadino all'esercizio dei diritti politici. E questi ultimi contraddistinguono l'evoluzione democratica dei Paesi occidentali sin dalle due rivoluzioni, quella francese e quella inglese. Ora, individuare nella stessa giornata i candidati che saranno scelti per rappresentare il nostro Paese nel Parlamento dell'Unione europea e negli organi di Governo delle autonomie locali

tra coloro i quali si siano candidati ad assumere la responsabilità di condurre le amministrazioni locali e degli enti locali. Certamente l'Italia e i Paesi dell'Unione europea

poi successivamente corroborate con la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha modificato la struttura elettiva delle Regioni nel nostro Paese, era quello di delineare un quadro di stabilizzazione politica degli amministratori locali,

sia comunale che provinciale, ed il presidente della Regione, sempre con la sua Giunta, essi rimangono in carica, e se si dovesse verificare una crisi, cade l'intera amministrazione comunale. Il brocardo, che ormai è invalso nel linguaggio giuridico-giornalistico, è appunto *simul stabunt, simul cadent*. Se noi proviamo a sottolineare questi passaggi così importanti, di certo non possiamo neppure sottacere il rilievo che poi era stato particolarmente esposto da alcuni emendamenti presentati in quest'Aula, ma che non ha potuto trovare accoglimento per il divieto che la legge n. 400 del 1988 pone in sede di conversione dei decreti-legge, cioè quello di far approvare proposte emendative in materia elettorale. Ebbene, noi avremmo dovuto affrontare il nodo della rieleggibilità dei sindaci dei Comuni sotto i 5.000 abitanti.

con la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato in radice il sistema del riparto legislativo tra Stato e Regioni,

che riguarda le autonomie locali, il sistema delle preferenze e anche tutto il sistema normativo possa essere oggetto di un raffronto con il sistema elettorale europeo.

e, quindi, in una condizione di particolare stress del sistema finanziario pubblico adotta delle misure particolarmente utili all'economia del nostro Paese, ma, soprattutto - ripeto - sarà oggetto di approfondimento e di riflessione proprio per mettere a confronto i due sistemi elettorali, il sistema degli organi di governo e delle amministrazioni delle autonomie locali e l'elezione del Parlamento europeo. europeo. Occorre anche sottolineare la particolare attenzione che il Parlamento nazionale dovrà

di governo in un Paese che ha una struttura federale e amministrativa ed in cui le Regioni esercitano una potestà legislativa e gli organi dei Comuni esercitano addirittura una particolare forma di autonomia che è prevista dagli Statuti. Sulla base degli studi più recenti e della migliore dottrina si sostiene persino che nell'esercizio dell'autonomia degli enti locali, che è stata individuata e descritta all'articolo 114 della Costituzione, si possa anche concretizzare un conflitto e quindi un'antinomia con le leggi dello Stato. Anche su questo terreno dovremo individuare un particolare criterio selettivo nell'esercizio delle potestà normative statutarie degli enti locali e legislative delle Regioni che a tutt'oggi non trovano evidentemente una struttura tesa a dirimere a dirimere questi conflitti nella Corte costituzionale.

cercato, in rapidissima rassegna, di sottolineare. Li supera semplicemente perché, individuando nella stessa giornata questo turno

in questa discussione generale hanno cercato di mettere in evidenza gli aspetti salienti e peculiari di un provvedimento che dà risposte ad un tipo di domanda che viene dalla gran parte dei nostri cittadini.

a recarsi più volte in un anno al seggio elettorale per poter esprimere le sue preferenze. Non è una cosa di poco conto negli ultimi anni abbiamo avuto un sensibile calo della percentuale della gente che si reca al seggio

questo, dal punto di vista della nostra democrazia così compiuta, non è un dato positivo. E allora - mi rivolgo a quelle istituzioni che non sempre sono vicine al cittadino quando si tratta di andare a votare il sindaco del proprio paese o della propria città si ha un contatto diretto: si conoscono i candidati sindaci e si va a votare sulla base della conoscenza della persona

evidenzia e apre un altro aspetto importante, che è quello del risparmio della spesa. Chi ha avuto la possibilità di amministrare un Comune sa bene quanti soldi

Noi siamo orientati all'espressione di un voto favorevole al provvedimento, che è stato illustrato con i dovuti approfondimenti dal relatore Malan

Qualche emendamento è stato anche presentato e io voglio ricordare, brevemente, quello riguardante la partecipazione degli osservatori alle elezioni europee a firma della nostra senatrice Rossana Boldi. Vedremo se esso troverà

senatore Boscetto.

ad alcuni emendamenti dichiarati improponibili per le ragioni che così bene ha spiegato il Presidente del Senato.

ha annunciato, come già prima di lui il ministro Maroni, che nella Carta delle autonomie andremo ad affrontare e risolvere qualcuno di questi temi, credo che la discussione in oggetto sia utile anche in questa sede. Porci i problemi serve per dare al Ministero dell'interno, al sottosegretario Davico e, prima di lui, al ministro Maroni qualche logica in relazione a queste problematiche. Qui noi troviamo l'emendamento 3.0.3, lo ribadisco - è stato dichiarato improponibile per le ragioni che ho spiegato (ma che tanto meglio di me ha spiegato il Presidente del Senato), dove si consente il terzo mandato consecutivo

o inferiore a 3.000 abitanti. Bisogna porsi il problema, in questo momento, con un puro intento speculativo, come dicevo

quindi l'inserimento di un terzo mandato per i sindaci di tutti questi Comuni avrebbe un peso notevole

con il ragionamento che in questi Comuni così piccoli il ricambio amministrativo è estremamente difficile. Pertanto, limitando a due mandati la possibilità per un buon sindaco di ricandidarsi, si provocano situazioni spesso negative, addirittura al limite del comico o del cattivo gusto.

ma sostituisce a se stesso persone che non hanno capacità amministrativa, che non sono in grado di reggere il confronto diretto che il sindaco deve avere con la società intesa nel senso più ampio. Quindi,

chi vuole abusare della situazione del proprio ente può farlo anche al primo mandato o al secondo, perciò la limitazione sta diventando, alla luce dell'esperienza,

Quello che poi non capisco - me lo spiegherà il collega Zanetta, tanto amico e tanto stimato - è come mai si voglia abolire il doppio turno per l'elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,

faticosi ed ovviamente raddoppiano i costi della consultazione elettorale. Le stesse ragioni che hanno dogmaticamente sorretto l'esigenza teorica del ballottaggio, alla luce della verifica fattuale negli anni, non hanno più particolari ragioni per esistere:

questa problematica mi stimola, anche perché sono stato presidente di Provincia, consigliere comunale, per cui ho vissuto queste problematiche settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. comunque il suo cordiale e cortese richiamo, sottolineando come questi pochi concetti che ho espresso - tante altre cose si potevano dire! - siano propedeutici a quella Carta delle autonomie

possibilmente distaccandoci dalle incrostazioni che si sono create nel tempo.

Saltamartini, Bodega e Boscetto per il contributo dato alla discussione: si tratta di un argomento importante di cui è bene studiare i dettagli. In particolare, il senatore Vita ha ricordato l'importanza di

particolare tipologia di provvedimento che affrontiamo, in particolare perché introducono temi che dovremo affrontare in futuro e che solo la particolare situazione nella quale ci troviamo ci impedisce di approfondire: ad esempio, le proposte dei senatori Gamba ed altri, Contini ed altri, che volevano rendere definitiva questa disciplina

i marittimi italiani all'estero tra coloro che possono esprimere il voto in quanto temporaneamente residenti all'estero. È necessità che era stata avanzata anche dal senatore Nespoli in Commissione: anche questo è un punto sul quale bisognerà tornare. Per intanto è importante varare il provvedimento all'esame, che comunque rappresenta, sia pure soltanto per questa scadenza, una importante agevolazione agevolazione a tutti per esprimere il proprio voto. se non la comunicazione al senatore Vita che tutta la problematica relativa all'informazione e pubblicizzazione delle elezioni per i cittadini neocomunitari è già in atto. Dal

parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 4 le parole: "senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" siano sostituite dalle altre: "senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva poi che, sebbene i nuovi oneri recati dal provvedimento siano coperti sul fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, ossia sul bilancio a legislazione vigente, tuttavia, il decreto-legge innova la legislazione vigente riducendo il periodo di apertura delle urne unificando così le modalità per tutti i tipi di elezione e determinando un sensibile risparmio. Sarebbe quindi più corretto, in occasione di analoghi provvedimenti, prevedere un meccanismo esplicito di compensazione tra i risparmi associati a modifiche legislative (quantificati nel dettaglio con la relazione tecnica) ed i nuovi oneri introdotti con il provvedimento. Per quanto concerne gli emendamenti, esprime parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 2.100, 2.0.103, 2.0.104 e 3.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché delle proposte 4.0.1 e 4.0.2, sulle quali il parere è di contrarietà semplice.". «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.300 (testo corretto) e 2.300 trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

la sottoscrizione delle liste dei candidati, il divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci, l'abolizione del doppio turno per l'elezione del presidente della Provincia, l'abolizione del doppio turno per l'elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i rimborsi elettorali relativi alle elezioni politiche, la revisione della disciplina generale del voto dei cittadini temporaneamente residenti all'estero. Pertanto, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono improponibili i seguenti emendamenti: 1.0.1,

millimetri del diametro dei contrassegni che vengono pubblicati sulleschede elettorali*.* Si tratta di una norma che è stata introdotta con la legge elettorale n. 270 del 2005per 2005per le elezioni nazionali, mentre per le elezioni europee vige ancora la vecchia norma, che riporta nell'Allegato B)

(come poi è stato fatto): se ne prevede l'inserimento nell'articolo 1, per cui si tratta di nuovo di una norma transitoria nell'ambito dei provvedimenti che vengono assunti per rendere possibile l'accorpamento delle elezioni e le particolari modalità

affrettato dal relatore - per cui le parole «le dimensioni dei» sono state soppresse e restano le parole «i contrassegni di tutte le liste di candidati

in quanto la modifica è inserita all'articolo 1 che, al primo comma, inizia con le parole «Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo

che, essendo inserita in questo comma, resta applicabile soltanto alle consultazioni di quest'anno. perplessità della Presidenza, con tutto il rispetto per la nostra attività legislativa, sull'opportunità di prevedere questa norma come transitoria e non come norma a regime. Forse,

potrebbe rendere un miglior servizio anche per il futuro. La mia è una semplice osservazione, visto che si sta ovviando giustamente ad un'anomalia, posta da alcuni colleghi, sulla differenza di dimensioni dei simboli tra elezioni politiche ed europee. In questo caso stiamo intervenendo soltanto per le elezioni europee, ravvisando comunque che l'anomalia esiste.

Si tratta di una norma che consentirà, se approvata, l'istituzione di un numero minore di sezioni per lo svolgimento

di conseguenza sarebbe possibile un notevole risparmio. Il Ministero dell'interno e il Ministero degli esteri sono stati consultati: entrambi ritengono fattibile questa innovazione, confermando che si tratterebbe di risparmiare una somma notevole. Credo pertanto che fosse opportuno presentarlo, sia pure fuori dai termini previsti per la presentazione degli emendamenti. Del resto, credo che la norma sia molto chiara.

per le elezioni politiche del 2008, hanno dato un'ottima prova e sono dunque state opportunamente riprese in questo decreto-legge con riferimento alle elezioni europee, con qualche ulteriore miglioramento opportunamente evidenziato dal relatore.

in un ambiente

tranquillamente a votare e pensa di esprimere il proprio consenso e quindi il suo consenso deve essere esaltato e tenuto in considerazione, credo che affrontare il tema dell'eliminazione del ballottaggio

semplicemente una norma richiesta dalla Commissione bilancio, per specificare che le misure previste nell'articolo stesso non devono comportare oneri. In sostanza, i funzionari che vanno a

avverto che le interrogazioni a risposta immediata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previste per la seduta pomeridiana di domani, concerneranno oltre agli argomenti già previsti, e cioè: condizioni di rischio sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria; privatizzazione della società Tirrenia e collegamenti con le isole minori,

soprattutto negli ultimi mesi, in cui siete venuti a Lampedusa a fomentare. Devo dare a qualcuno la responsabilità di tutto quanto è successo.

il nostro vivo dispiacere per l'incendio che si è sviluppato nel centro e anche noi esprimiamo piena solidarietà alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco che si sono adoperati in un contesto difficile

il ruolo che abbiamo assegnato a Lampedusa possa essere condiviso da tutti. C'è bisogno di una profonda revisione della funzione che abbiamo assegnato a quella piccola isola. È sbagliato

corso diverse proteste, anche clamorose, come quella del consiglio comunale di Lipari che si trasferisce a Sanremo per protestare contro i tagli alla Siremar.

all'interrogazione, in modo tale che insieme si possa trovare la migliore soluzione, una soluzione che possa essere corrispondente a quello che le comunità delle isole minori richiedono a tutti noi.